il disegno di legge contenente norme sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche a nostro avviso è ancora una

i cosiddetti decreti legislativi, ma sulla base e con l'osservanza di «principi e criteri direttivi» molto chiari e omogenei e soprattutto molto stringenti e dettagliati, definiti dal Parlamento. In una legge delega la mancanza o l'indeterminatezza di tali principi e criteri direttivi comporta che l'unico criterio direttivo per la normazione dell'oggetto della delega sarebbe quindi il libero apprezzamento del Governo e proprio un simile assetto è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale dell'8 ottobre 2007, n. 340.

Mancano infatti - in molteplici oggetti - indicazioni dì contenuto sufficienti a circoscrivere la discrezionalità del legislatore delegato.

In particolare, all'articolo 9 è difficile ipotizzare quanti decreti legislativi saranno necessari per i ruoli unici, con annesse tre procedure e quattro mesi di tempo. Si tratta, in una parola, di una delega che prevede tempi molto lunghi e di incerta determinazione. Per quanto concerne il principio afferente alla «determinazione di principi e criteri direttivi relativi ad oggetti definiti» gli articoli 2, 4 e 7 riportano disposizioni contenenti principi e criteri generici. Inoltre, il progetto governativo è caratterizzato, in molte sue parti, da una forte tendenza iperaccentratrice nelle mani del solo Presidente del Consiglio, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 5 della Costituzione, che definisce il nostro modello organizzativo fondandolo sul più ampio decentramento amministrativo amministrativo nell'attuazione dei servizi basato su un forte carattere di autonomia. Il comma 3 dell'articolo 3 estende in modo generalizzato il meccanismo del silenzio assenso anche nei procedimenti «in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini». Fino ad ora il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 241 del 1990 esclude il silenzio assenso per i procedimenti aventi ad oggetto interessi sensibili, nel presupposto - costituzionalmente ineccepibile, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale - di una prevalenza del pubblico interesse su quello dei privati cittadini in casi in cui sono coinvolti interessi di rango costituzionale, come nei casi del patrimonio culturale e dell'ambiente ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione: «Nella materia ambientale vige un principio fondamentale, ricavabile da una serie di disposizioni, da interpretarsi unitariamente nel sistema, secondo cui il silenzio dell'amministrazione preposta al vincolo ambientale non può avere valore di assenso» (sentenza n. 26 del 1996 e n. 440 del 1997). La previsione, contenuta nell'articolo 7, comma 1, lettera *a*), dell'assorbimento di uomini, mezzi, esperienze e capacità affermate in anni di impegno nella difesa dell'ambiente, del territorio

e necessarie per il rispetto dei principi sanciti dall'articolo 9 nell'eccezione più ampia della tutela dell'ambiente e del territorio; Ministri"; all'articolo 9, comma 1, lettera *b)*, numeri 2 e 3, si estende il ruolo unico anche ai dirigenti delle Regioni e degli enti locali, incidendo sulla materia riguardante l'organizzazione degli uffici che l'attuale articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza esclusiva delle singole Regioni. Inoltre, la previsione contenuta al comma 1, lettera *g)*, dell'articolo 9, secondo la quale la quale il dirigente pubblico privo di incarico, dopo un determinato periodo di collocamento in disponibilità, decade dal ruolo unico, configura un vero e proprio licenziamento. L'assenza di incarico non può essere attribuita solamente alla responsabilità del singolo dirigente,

dal comma secondo dell'articolo 97, che garantisce un'organizzazione dei pubblici uffici tale da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Inoltre, i dati e gli elementi riportati nella relazione tecnica non danno la necessaria garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in presenza della clausola di invarianza prevista dall'articolo 16 e della norma di salvaguardia prevista dall'articolo 17. Per tutti questi motivi, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge. Salutiamo gli studenti e i docenti dell'Istituto comprensivo «Alcide De Gasperi» di Castello di Cisterna, in provincia di Napoli, che stanno seguendo i nostri lavori.

i colleghi che mi hanno preceduto hanno già ampiamente illustrato il senso del provvedimento in oggetto: si tratta di un disegno di legge che segue il decreto-legge il decreto-legge n. 90 del 2014, ancora legato al riordino della pubblica amministrazione, che noi reputiamo giusto negli obiettivi, ma assolutamente inefficace nei risultati ed inopportuno nel metodo. Vorrei dire una parola di ringraziamento al Ministro, che è stato presente in Commissione per operare quella dialettica parlamentare che purtroppo si potrà celebrare forse solo in quella sede, vorrei ringraziare il Sottosegretario, che ugualmente ha seguito i lavori, e vorrei ringraziare il relatore, che è stato parte così significativa ed importante di questo provvedimento. Purtroppo infatti, fermi i ringraziamenti al Governo e al relatore, la *magna pars* delle modifiche che sono state attuate in 1a Commissione nasce da emendamenti del relatore e questo non è casuale, ma è estremamente significativo, perché purtroppo dà la misura di come questo sia un provvedimento *monstre*, un provvedimento *omnibus*, come lo ha giustamente definito il senatore Candiani, che tratta temi sconfinati, che contiene deleghe oceaniche, che presuppone decreti delegati numerosissimi. Stiamo parlando di un provvedimento che si è munito di un paio di articoli in più in Commissione, quindi di un provvedimento che si compone di quattro capi e di 17 articoli, con con una media di quattro articoli per capo, che contiene dieci deleghe al Governo su temi di significato capitale, inerenti alla pubblica amministrazione, alla semplificazione normativa e regolamentare, al riordino dei servizi pubblici locali, alla riorganizzazione delle partecipazioni pubbliche detenute dalle pubbliche amministrazioni, all'impiego pubblico, alla dirigenza pubblica, al riordino dei corpi di Polizia, alla segnalazione certificata di inizio attività ed al silenzio assenso ad essa connesso, alla Conferenza di servizi. Colleghi, si tratta di argomenti immensi, vastissimi nella loro complessità, che avrebbero meritato, *in primis*, un alveo parlamentare più significativo e secondariamente ciascuno di questi argomenti avrebbe meritato una delega a sé, avrebbe meritato una trattazione, un disegno di legge a sé, necessario e sufficiente per approfondire con la dovuta serietà ed efficienza - lo sottolineo - materie di importanza così capitale, per rispondere ad una domanda alla quale ormai non ci possiamo più sottrarre. E io, ministro Madia, la ringrazio ancora una volta, perché comprendo la sua presenza in Commissione non è banale, né scontata; lei è l'unico Ministro che l'abbia fatto. Però, signora Ministro, voi avete scoccato la freccia, ma non avete centrato il bersaglio. Dalla relazione illustrativa risulta che il primo obiettivo è quello della riduzione dei costi della pubblica amministrazione. Signora Ministra, lei sa benissimo - perché ce l'ha detto la Corte dei conti in audizione, ce l'ha detto la Banca d'Italia, ce l'hanno detto le associazioni di imprenditori e di consumatori, ce l'ha detto, a livello internazionale,

per cento di riduzione della spesa del corpo centrale dello Stato comporterebbe un aumento dello 0,9-1 per cento del prodotto interno lordo ed un conseguente aumento dell'occupazione. Il provvedimento in esame anzi ci sarà un carico di costi, derivante dall'accorpamento, dalla riorganizzazione, dalla riruolizzazione di dirigenti e forze di polizia. È ben vero che esiste una clausola di invarianza, ma purtroppo ormai questa è diventata una clausola di stile. Si dice che queste più di quello che è previsto dalle coperture del provvedimento. Signora Ministro, non è vero, tanto che l'articolo 17 dice che, ove vi fossero nei decreti delegati dei costi in più, i provvedimenti contenuti nei decreti delegati stessi si rimanderebbero. colleghi, questa non è una soluzione: questo è un rinvio, questa è una politica dello struzzo. Ancora: uno degli obiettivi è la riduzione della complessità (questo dice la relazione illustrativa a questo provvedimento). Come sappiamo - consentitemi una citazione kafkiana le catene delle imprese e quindi dei cittadini utenti stanno nelle carte dei regolamenti inutili. Purtroppo, colleghi, i regolamenti inutili non sono stati eliminati da questo provvedimento. Ci sono 400 decreti delegati, ereditati dai Governi precedenti, ma anche creati da questo Governo, che attendono un'attuazione. Ci sono purtroppo ulteriori deleghe contenute in questo provvedimento, che non sarà facilissimo attuare, anche sotto il profilo temporale.

sono principi e criteri direttivi di cui non si comprende il senso e che si prestano purtroppo ad interpretazioni costituzionalmente irragionevoli.

alcuni accenni al contenuto; a questo proposito, vorrei fare un ampio rimando al testo scritto della nostra questione pregiudiziale. Alcuni temi sono già stati toccati dai colleghi che mi hanno preceduto e si tratta di temi capitali. Quando parlo di disomogeneità delle deleghe, colleghi, mi riferisco a contenuti e a provvedimenti, all'interno di questo disegno di legge, che coprono materie già normate da provvedimenti precedenti. Un esempio? L'autotutela amministrativa, la segnalazione certificata di inizio attività e il silenzio-assenso, che sono già stati normati con il decreto‑legge in tema di grandi opere, apertura dei cantieri e velocizzazione delle opere nel nostro Paese, nel 2014. Un altro esempio? Sull'indipendenza, imparzialità e trasparenza dell'azione della pubblica amministrazione esiste un decreto legislativo del 2013, che copre i temi di inconferibilità ed incandidabilità che vengono trattati in questo provvedimento. E purtroppo, colleghi, per il problema della successione delle leggi nel tempo, che non è così automatica (noi lo sappiamo), c'è una sovrapposizione incongrua e casuale

altri esempi di natura marcatamente politica. Noi ormai siamo schiavi della dittatura del messaggio accattivante. Si è detto che è stato abolito o drasticamente ridotto il Corpo forestale. Come ricordava la collega De Petris, siamo sicuri che di questo ci dobbiamo compiacere? Ancora una volta, faccio riferimento all'opacità e alla mancanza di coordinamento con disposizioni precedenti

Qual è il messaggio che passa da una considerazione di questo tipo? C'è chi vuole abolire i forestali ottenendo un risparmio di spesa, che peraltro non si realizza, colleghi: ci costerà, infatti, di più

vorrei ricordare l'articolo 9, ex articolo 10 sulla dirigenza pubblica. Al netto della inspiegabile eliminazione - non esiste una *ratio* e anche questo lo trovo costituzionalmente illogico - della figura del segretario comunale, vorrei capire per quale motivo il ruolo unico di tre livelli di Governo e di Governo e di dirigenza pubblica, oltre che di professionalità, dovrebbe portare un beneficio all'imparzialità, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione: porterà ad una confusione di competenze, ad una mobilità spesso inefficace. Per quale motivo dovrebbe diventare un migliore direttore generale di un Ministero un dirigente comunale anziché un dirigente dell'amministrazione centrale che è stato formato esattamente per essere un dirigente generale ministeriale?

che, ancora una volta, siamo di fronte a un gioco delle parti, senz'altro reso gradevole dagli interventi appassionati dalla senatrice Bernini, capace di mettere una passione francamente ammirevole su delle battaglie che meriterebbero una diversa passione. Nulla è più stucchevole che questa ennesima discussione sulle pregiudiziali di costituzionalità di norme che sono state ampiamente dibattute, discusse, esaminate e sviscerate all'interno della Commissione. Tali norme hanno visto un concorso del Parlamento, riconosciuto da tutte le parti

la Commissione, non soltanto ha proceduto ad una amplissima indagine conoscitiva audendo un numero elevatissimo di esperti esperti e persone coinvolte direttamente nell'amministrazione, di responsabili, di enti e di organi che vengono interessati da questo provvedimento. Dunque, la Commissione ha ampiamente dibattuto nel merito e ha avuto la possibilità di

hanno avuto modo di essere ampiamente schiariti. C'è stato un concorso corale da parte di tutti i Gruppi, sia in fase di discussione generale all'interno della Commissione sia in fase di dibattito sugli emendamenti. il provvedimento è stato profondamente cambiato e mutato. È un provvedimento assolutamente virtuoso dal punto di vista dell'approfondimento del dibattito di merito, anche in relazione alle pregiudiziali di costituzionalità: ne è prova la genericità con la quale oggi vengono presentate tali questioni pregiudiziali, buttate lì tanto per metterle avanti, come per non lasciare nulla di intentato, anche se, francamente, sono del tutto inconsistenti nel merito.

del mantenimento o della ristrutturazione del Corpo forestale dello Stato. A questo proposito, mi permetto di ricordare fin da ora che l'Italia è l'unico Paese in Europa ad avere un Corpo forestale dello Stato. Dubito che gli altri Paesi europei di lunga tradizione costituzionale debbano essere considerati incostituzionali loro stessi perché non hanno il Corpo forestale dello Stato. sia fragile in questo momento la critica portata a questo provvedimento. In realtà, questo è un provvedimento di grande portata, che incide profondamente sulla futura organizzazione della nostra vita amministrativa.

che vengano predisposti dei criteri di delega, che sono in questo caso assai specifici (anche per effetto del lungo dibattito svoltosi in Commissione), e che sia poi il Governo a procedere ai decreti attuativi di queste deleghe, sapendo che in futuro, comunque, ci sarà ancora tempo per il Parlamento per esprimersi sull'attuazione di questi decreti attuativi.

alla sentenza della Corte costituzionale (che nulla dice di più rispetto a quanto già sappiamo), che vengono ritualmente reiterati e rievocati come se fossero delle eccezioni in qualche modo pertinenti. Ma cosa vuol dire che il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o a criterio direttivo in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, qual è per definizione la legislazione su delega? la consistenza di questo provvedimento all'esame dell'Assemblea sia sufficientemente specifico e preveda questi criteri e questi principi. Dunque, tutto si può dire tranne che sia delegato soltanto al libero apprezzamento del legislatore l'esercizio dei criteri di delega. Affermare questo significa non avere forse neanche letto fino in fondo e non avere compreso pienamente il provvedimento.

pretendere una legittimità costituzionale su un atto che nasce per iniziativa del Governo ed è stato da questo definito in termini di ciò che si poteva o non si poteva approvare in Commissione. Abbiamo avuto solo emendamenti del relatore, con qualche rara eccezione, peraltro

13 (ex 14), che aveva a che fare con le partecipazioni azionarie detenute dai Comuni e dalle amministrazioni pubbliche e con i servizi pubblici erogati.

interesse privato, tra i fini della pubblica amministrazione, e cioè la gestione dei servizi per i cittadini al minor costo e con la miglior qualità, rispetto al fine di lucro perseguito, pur legittimamente, dai privati ma nel mercato e nel settore privato. semplicemente un gesto di coerenza ed invece si è adottata, nel testo del relatore, una formula volutamente ambigua, che antepone la legislazione europea rispetto a quella italiana, disconoscendo che i *referendum* del 2011 avevano avuto piena legittimazione anche rispetto

del Senato in questo caso, ma in generale del Parlamento, decidendo ciò che si può e ciò che si vuole. Arriviamo quindi a due paradossi.

Il Governo vede il Parlamento come un agente di disturbo e non di controllo, non come il titolare della funzione legislativa, ma come un impiccio sulla strada

stanno portando a casa ciò che volevano, vale a dire la rimozione del Corpo forestale dello Stato, unica forza peraltro toccata da questo provvedimento, che puntava all'armonizzazione e alla sintesi tra cinque forze dell'ordine diverse. Ebbene, ne hanno toccata solo una, quella che - guarda caso - è il baluardo rispetto ai delitti ambientali, delitti ambientali, la più efficiente e più libera rispetto al potere politico, rispetto ad altri organi di controllo locali spesso lottizzati e asserviti. Noi non possiamo fidarci, non possiamo dare a questo Governo il nostro silenzio assenso. Per questo sono state presentate delle questioni pregiudiziali e non riteniamo di dover procedere all'esame

abrogare le norme che prevedevano decreti attuativi a partire dalla fine del 2011. Dobbiamo sapere che, con questa delega, diamo al Governo la possibilità

a cosa ottemperare e cosa ignorare, andando a tagliare e a ricucire tutto quello che oggi diciamo. Noi questa delega in bianco al signor Renzi e ai suoi manovratori non la possiamo dare.

quando pensa di poter intervenire in maniera incisiva su una macchina importante e complessa come quella dello Stato. Tuttavia, il problema che noi ci siamo posti - è già stato detto anche nella discussione sulle questioni

che il Parlamento dà al Governo su una serie di materie centrali e importanti che avrebbero avuto bisogno perlomeno di una discussione

Vorrei dire ai colleghi parlamentari, se ancora pensano di avere una loro portata legislativa, che qui riusciamo a fare addirittura una cosa al contrario, che può essere poco importante, se volete, dall'esterno. Noi riusciamo persino a dare la delega al Governo per definire, in relazione alle esigenze connesse, il diritto dei membri del Parlamento:

continuità del lavoro svolto dalla Guardia forestale, asserendo che, proprio in un momento in cui ci sono particolari percezioni sulla delicatezza dell'ambiente, si vuole smantellare l'unica forza che probabilmente ha le competenze specifiche continuative per lavorarci.

cui si sentono brutte storie. O si sceglie di mettere figure di garanzia, come potevano essere i segretari comunali, addirittura dandogli poteri più ampi, o si

che - ad esempio - si occupano di energia di mestiere e noi mettiamo nelle loro mani la delega su aziende che trattano anche di energia. Mi permetta una battuta: battuta: è come mettere Dracula alla Presidenza dell'AVIS. *(Applausi dal Gruppo LN-Aut)*. Visto quello che è successo con le banche e con altre cose, forse un minimo di riflessione tutti insieme dovremmo fare. Credo che l'interesse comune delle aziende che lavorano sul territorio debba essere stralciato e trattato in maniera autonoma.

Il Governo Renzi, in realtà, aveva altre intenzioni ed era partito con l'ipotesi di accorpamenti ben più ampi delle forze di polizia: che vi sia quest'intenzione nell'azione del Governo l'ha confermato qualche giorno fa il vice ministro Morando - persona che ben conosciamo qui al Senato che non parla a caso - il quale in un'intervista ha detto che le forze di polizia dovrebbero essere una sola o, al massimo, due. Ora, che si discuta da anni di accorpamenti e razionalizzazioni è un dato di fatto, questo sia utile al Paese è tutto da dimostrare. Probabilmente, se colonizzassimo un nuovo pianeta e sbarcassimo tutti su Marte, iniziando da zero una nuova era,

C'è, insomma, un vissuto della nostra Nazione che non può essere cancellato ed eventuali interventi di razionalizzazione comporterebbero più problemi e costi che soluzioni.

che interventi di più ampia portata. Renzi, così, potrà dire: «Abbiamo ridotto le forze di polizia, che non sono più cinque, ma quattro!». Forse non sa neanche quali siano o cosa facciano, ma l'importante è raccontare qualcosa.

poi dei problemi nell'accorpamento del Corpo forestale dello Stato con la Polizia, sotto vari profili. In primo luogo, non sarebbe possibile proseguire nella gestione delle 150 riserve naturali statali, costruite su terreni demaniali, assicurata oggi, a costi molto contenuti, anche da personale gestito personale gestito dal Corpo forestale dello Stato, in virtù di specifiche norme. Ci sarebbero duplicazioni di strutture tra Carabinieri e Polizia di Stato, e quest'ultima dovrebbe gestire

i servizi e i corpi di polizia provinciali, che operano a livello locale, a fronte di un corpo di polizia che opera a livello nazionale. Per quanto riguarda poi le attività delle Province, faccio presente che si pone un problema. Con la presunta abolizione delle Province resta il problema delle polizie provinciali che, essendo in genere addette a compiti relativi

per quanto riguarda il rischio idrogeologico, i censimenti naturalistici, l'educazione ambientale e tante altre questioni. Nei giorni scorsi, il comandante del Corpo forestale dello Stato della Campania ha ricordato - ad esempio - un tema che, nell'Aula del Senato, viene spesso evocato, ovvero la terra dei fuochi

anche quando, in televisione, *fiction* ispirate a questo tipo di impegno raggiungono vette di ascolto superiori ai normali prodotti

caos, confusione e sovrapposizioni, mentre altro è andare a determinare con più precisione le competenze delle singole forze di polizia. Questo sì, si può e si deve fare per garantire risparmio. Se la Polizia di Stato è specializzata nel campo della comunicazione perché ha sviluppato, attraverso l'evoluzione della

generale, abbiamo nuclei che svolgono attività similari e determinano sprechi e sovrapposizioni. In tali casi si può intervenire, razionalizzando ed evitando intrecci ma non certo aggredendo il Corpo forestale dello Stato, nei confronti del quale gli italiani hanno stima, il quale svolge un compito rilevantissimo e oggi, di fronte all'accresciuta sensibilità ambientale e alla maggiore preoccupazione per la tutela del territorio, è chiamato a esercitare funzioni indispensabili. Noi, nel sostenere i nostri emendamenti, siamo certi che in Aula si potrà generare un consenso virtuoso, positivo e trasversale per evitare, tra i tanti errori, che venga commesso anche questo all'interno di un demagogico, inefficace e solo dannoso riordino presunto

intervengo in discussione generale su questo disegno di legge per la riforma della pubblica amministrazione segnalando che esso ci offre la possibilità di intervenire nell'ambito molto particolare della ricerca in università e, in particolare, negli enti pubblici di ricerca.

al mondo della ricerca rispetto alla pubblica amministrazione. L'assimilazione degli enti pubblici di ricerca nella pubblica amministrazione, comporta una serie di problematiche che mal si adatta al lavoro di ricercatore. Ricordo che la figura del ricercatore è molto particolare ed ha caratteristiche che non si riscontrano in altre figure professionali della pubblica amministrazione. Il ricercatore gode - ad esempio - della libertà di ricerca e dell'autonomia professionale, che deriva direttamente dalla Carta europea dei ricercatori, che l'Italia ha recepito. Il suo è un lavoro profondamente intellettuale, che non trova riscontro in altri settori. Eppure, si pensi che in questo momento un architetto dell'ufficio del catasto è trattato alla stessa stregua, dal punto di vista normativo, di un ricercatore di un ente pubblico di ricerca.

D'altronde, l'articolo 33 della Costituzione recita che le arti e la scienza sono libere e libero ne è anche l'insegnamento. Pertanto, questa eccezione culturale scaturisce direttamente dal dettato costituzionale.

pubblici di ricerca; uno statuto speciale per la ricerca, che la scorpori dal resto della pubblica amministrazione, e, infine, una contrattazione in comparto separato per i ricercatori e i tecnologi degli enti pubblici di ricerca.

pensi - ad esempio - alle normative sulle missioni o sul *turnover*: gli enti pubblici di ricerca hanno sofferto, in passato, delle limitazioni sul *turnover*, che sono derivate direttamente da quelle imposte alla pubblica amministrazione ed hanno causato una progressiva riduzione del numero dei ricercatori impiegati in enti pubblici di ricerca. ricerca. Un comparto separato, pertanto, darebbe la possibilità di operare attraverso quel principio di autonomia responsabile,

Si richiede, quindi, la possibilità di intervenire, anche con le assunzioni e le progressioni di carriera svincolate dalle limitazioni del *turnover*, in piena autonomia e con valutazioni *ex post*

perché vige l'equiparazione al resto della pubblica amministrazione, che non è consona al funzionamento degli enti pubblici di ricerca. Chiedo, quindi, al Governo e al relatore la possibilità di riflettere su

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, giunge in Aula un provvedimento che l'Italia attende da tempo e che è cruciale per la modernizzazione del Paese. La riforma della pubblica amministrazione è stata ripetutamente indicata come una misura decisiva, ma è stata spesso invocata con spirito benaltrista rispetto alle varie riforme che la classe politica ha intrapreso. Questo atteggiamento non ha fatto difetto nemmeno in occasione delle riforme costituzionali e della legge n. 56, che ha dato seguito alla formazione delle Città metropolitane. Ma la spinta riformatrice che il Governo Renzi ha messo in campo non si è fermata e non solo ha proposto azioni immediate a fronte di problematiche urgenti con il decreto Madia, ma ha anche rilanciato un coordinato insieme di norme e deleghe che non è eccessivo dire che rivoluzioneranno la pubblica amministrazione. Vedete, colleghi, non è irrilevante sottolineare questo fatto: stiamo riformando lo Stato italiano nelle sue varie articolazioni e livelli. Lo stiamo modernizzando, e ciò significa che stiamo cercando di renderlo fattore di competitività, e non più freno alla piena espressione delle potenzialità dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Su questo punto voglio fare relativa ad un incontro pubblico che, da giovane segretario comunale del Partito Popolare, organizzai in occasione della campagna elettorale del 1996, quando era candidato al Senato, nel collegio del mio territorio, il professor Andrea Manzella, il quale mi propose di invitare Beniamino Andreatta. Lo andai a prendere a Bologna e, durante il viaggio, avemmo modo di parlare - guarda caso - della pubblica amministrazione, tema che egli riprese durante il suo discorso al pubblico, facendo un esempio. Se chiediamo ad un funzionario della pubblica amministrazione francese di descrivere sinteticamente il suo lavoro, ci sentiremo rispondere che consiste nell'aiutare lo sviluppo del proprio Paese. Se rivolgiamo la stessa domanda ad un funzionario tedesco, ci sentiremo rispondere che consiste nel facilitare la vita di cittadini e imprese. Se poniamo la domanda ad un funzionario italiano, ci dirà che lui sta lì per far rispettare la legge.

leggi. Una parte importante della sfida viene raccolta con il disegno di legge in esame, di cui cito solamente gli articoli 2, 3 e 4, riguardanti la Conferenza di servizi, il silenzio assenso e il riordino dei regimi autorizzativi, sottolineando la decisività dell'attuazione dell'articolo 1 sulla cittadinanza digitale, che diventa il principale di criterio ordinatore della nuova pubblica amministrazione. In secondo luogo, modernizzare lo Stato significa che stiamo cercando di renderlo fattore di omogeneità nel Paese, e non di differenze. Su questo punto voglio soffermarmi, perché lo ritengo un aspetto tenuto troppo sotto traccia. Le forbici che dividono il Paese sono tante, ma non possiamo permetterci più che fattore di queste differenze sia la disomogeneità della pubblica amministrazione. Lo dico sapendo che provengo da una Regione, l'Emilia-Romagna, che a ragione è spesso guardata come riferimento per procedure, organizzazione, capacità di controllo e di programmazione della spesa. Ma anche in Emilia-Romagna abbiamo consapevolezza di due cose. La prima, che tra l'altro il nuovo presidente Bonaccini ha messo in testa al suo programma, è la semplificazione normativa. La seconda è la partecipazione ad un comune impegno per rendere omogeneo il Paese, che non può vedere territori "in fuga" attraverso procedure avanzatissime, perché le forbici si aprono con il movimento di tutte e due le lame. Faccio un esempio molto chiaro: l'introduzione della TARI è avvenuta nel momento in cui era concluso da tempo, per buona parte dei Comuni dell'Emilia-Romagna, il passaggio da tassa a tariffa. Molti Comuni avevano già smantellato gli uffici di riscossione della tassa rifiuti e del recupero di morosità connesso, perché centinaia di migliaia di cittadini pagavano già la bolletta al gestore del servizio. Oggi li hanno dovuti riattrezzare, dovendo gestire anche gli sbilanci finanziari tra quanto devono versare al gestore del servizio e quanto riscuotono con la TARI. Siamo tornati indietro. Almeno io la penso così, anche se devo riconoscere che in Italia non si può mai essere sicuri se il senso che stiamo percorrendo sia l'avanti o l'indietro. amministrazione deve fare questo: stabilire nel breve, nel medio e nel lungo periodo il senso dell'andare avanti. Per concludere questo inciso, voglio mettere in rilievo la riforma Boschi del Senato, che stiamo portando avanti nei due rami del Parlamento. Il Senato delle Regioni va visto anche come una grande opportunità

che il Senato riformato, nella sua nuova composizione, renderà possibile. In terzo luogo, modernizzare lo Stato significa cercare di renderlo adeguato a tutti i livelli istituzionali e amministrativi ai suoi essenziali compiti di azione, tutela e garanzia, evitando di vederlo disordinatamente presente in troppi ambiti che non gli competono. Questo è un tema cruciale se si vuole dare un senso alla ricorrente discussione sul ridimensionamento della spesa pubblica. In conclusione, vorrei intervenire brevemente sulle società partecipate di gestione dei servizi pubblici locali. Se in una prima fase storica la creazione di società strumentali con l'esternalizzazione dei servizi ha avuto il merito di identificare la dimensione di centri di costo che non erano riconoscibili all'interno dei bilanci comunali, la successiva normativa ha sviluppato con sufficiente coerenza una visione sostanzialmente industriale, basata sulla convinzione che le reti infrastrutturali sono fattore decisivo della competitività di un territorio. un territorio. Le reti infrastrutturali e gli *asset* sono detenuti dai territori, ma sono gestiti imprenditorialmente e l'efficienza della gestione imprenditoriale si verifica solo con quel *check point* che è la messa a gara dei servizi. Gli enti locali controllano l'adeguatezza dei costi del servizio anche in relazione agli investimenti che sviluppano e mantengono l'efficienza delle reti. Anche qui mi rendo conto di avere alle spalle un territorio, quello emiliano romagnolo, dove i Comuni, centinaia di Comuni, hanno condiviso una scelta strategica. La storica presenza delle società municipalizzate ha rappresentato un importante patrimonio di competenze tecniche e umane, di investimenti delle comunità locali, che nei decenni hanno reso pari opportunità ai cittadini, ma soprattutto hanno reso possibile un grande livello di sostenibilità del nostro sviluppo, anche quando il concetto non era così diffuso nella coscienza dei cittadini. efficientare le aziende, riorganizzarle, dare loro massa critica, costituire economie di scala che ci dessero la possibilità di vincere le gare e continuare a gestire con le nostre società i servizi pubblici locali, proprio per non svendere tutto quel patrimonio formato in decenni che proprio con questa scelta aveva la grande possibilità di essere non solo adeguato nella somministrazione dei servizi, ma poteva restituire risorse alle comunità.

Ministro, colleghi, il disegno di legge oggi in discussione parte dalla condivisibile necessità di razionalizzare e semplificare il funzionamento della pubblica amministrazione, al fine del raggiungimento di due, altrettanto condivisibili, obiettivi: garantire garantire un più efficace funzionamento interno delle pubbliche amministrazioni ed assicurare un'erogazione più rapida e trasparente dei servizi al cittadino. Leggendo però i contenuti del disegno di legge, ci si accorge di quanto siano, come dire, «originali e controverse» le misure con le quali il Governo intende rispondere alla richiesta, peraltro legittima, da parte della collettività, di maggior efficacia e professionalità nella somministrazione delle prestazioni. Ascoltando i colleghi che mi hanno preceduto e lo stesso senatore Gasparri, mi preme rilevare che una delle criticità contenute nel provvedimento è senza dubbio la soppressione del Corpo forestale dello Stato e il suo assorbimento alla Polizia di Stato. È una decisione incomprensibile, che lascia francamente basiti, visto che contribuisce al depauperamento di tutte quelle attività di controllo del territorio, tipicamente messe in atto dai forestali e finalizzate alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica. La scelta del Governo di eliminare il Corpo forestale dello Stato è, infatti, ingiustificabile, a fronte dell'altissima specificità e professionalità che contraddistingue l'attività di polizia ambientale svolta da quest'ultimo, competenze enormi che hanno permesso, soprattutto negli ultimi anni, l'accertamento di gravissimi reati contro il territorio e l'ambiente. Due esempi valgono su tutti: la terra dei fuochi e la mega discarica abusiva di Bussi, scoperta proprio dalla Guardia forestale nel 2007. Il Movimento 5 Stelle è totalmente contrario alla sua soppressione e lo abbiamo abbondantemente dimostrato anche nel corso di una conferenza stampa, nonché presentando in Commissione diversi emendamenti, tutti respinti, e che, alla luce della manifestazione che si è tenuta solennemente martedì scorso, ci auguriamo vengano presi in considerazione in Aula da un Governo che fa della superficialità e del pressappochismo il *dominus* della sua azione. Un altro aspetto che impone sicuramente una riflessione è quello relativo alla delega al Governo in materia di conferenza dei servizi, soprattutto nel passaggio del testo in cui si prevede che «si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni che, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbiano espresso, nelle forme di legge, la propria volontà, e questo, anche se siano amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente». La progressiva e documentata permeabilità della pubblica amministrazione ai fenomeni di corruzione impone una seria riflessione sull'effettiva utilità di una norma che, se approvata, produrrebbe un ulteriore assalto alla diligenza da parte di organizzazioni criminali tradizionali e centri occulti di potere o affaristici che, in nome del profitto (e solo del profitto), e mettendo in campo un'ineguagliabile incoscienza e spregiudicatezza, potrebbero essere facilmente autorizzate autorizzate all'utilizzo, per meri fini privatistici e di *business*, di beni dall'inestimabile valore ambientale, storico e artistico. Chiedo che su questo venga fatta attenzione attenzione e venga seriamente posto un freno alla corruzione. Consentitemi, poi, di soffermarmi sulla delega contenuta nell'articolo 9 del disegno di legge, riguardante la dirigenza pubblica e la valutazione dei rendimenti di tutti i pubblici uffici; un punto del provvedimento sul quale il Governo dimostra tutta la sua confusione in merito alle funzioni e allo *status* della dirigenza scolastica. La delega in questione prevede che venga istituito un ruolo unico presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in cui confluiscono i dirigenti delle università statali, degli enti pubblici di ricerca, delle Camere di commercio e vengono esclusi, a causa della natura non gestionale del proprio ruolo, i dirigenti scolastici. Tuttavia, nel Tuttavia, nel disegno di legge definito impropriamente dal Governo «la buona scuola», si riconoscono ai dirigenti scolastici incarichi di natura prettamente gestionale e manageriale, riconoscendo a questi ultimi, oltre al potere di scegliere la propria squadra di docenti, con chiamate dirette, anche la possibilità di individuare percorsi formativi e di valorizzazione del merito scolastico alternativi a quelli tradizionali, mediante l'ottenimento di finanziamenti esterni e sponsorizzazioni. È chiaro, pertanto, che il Governo ha volontariamente deciso di depotenziare la funzione pubblica pubblica del dirigente scolastico, facendo venir meno la sua specificità e il suo ruolo di buon padre di famiglia nella programmazione e svolgimento delle attività didattico-creative, decidendo di trasformarlo in un capo d'azienda, prevalentemente vincolato ad una fredda analisi costi-benefici nella realizzazione della sua *mission* educativa, senza che dal 2000 sia stata portata avanti una seria preparazione di dirigenti e *manager*

in questo modo, o per il delfinario a Rimini o per interventi a gamba tesa in varie parti d'Italia, la Forestale rischia di non essere più l'amica, la consulente sul territorio, specialmente nelle zone più disagiate di montagna,

debba essere utilizzato per dare un contributo migliore ad una riforma che ha una funzione fondamentale, un ruolo centrale nel vasto programma di riforme che il Governo e la maggioranza stanno portando avanti in relazione

Credo corra l'obbligo di ringraziare innanzitutto il Governo, per il coraggio e la determinazione nel portare avanti questa riforma, che potremmo definire la riforma delle riforme per la funzione e l'importanza che riveste la pubblica amministrazione e per il livello di inefficienza ed inadeguatezza, seppure con le dovute eccezioni, che oggi essa rappresenta in termini reali e nel sentimento del nostro Paese. Un ringraziamento particolare va alla Commissione ed al relatore, che hanno dato un contributo importante per migliorare il testo del Governo. Governo. Che cosa hanno in comune il Ministero dell'interno, il Comune di Milano, l'Istituto nazionale di previdenza sociale o l'Istituto autonomo case popolari di Trapani? Sono organizzazioni legate tra loro da uno scopo comune, ovvero quello di consentire alla nostra Repubblica di raggiungere i suoi obiettivi costituzionalmente individuati quali il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica (il Ministero dell'interno), la raccolta di contributi e l'erogazione di prestazioni sociali (l'INPS), la realizzazione di case popolari e la loro assegnazione a persone non abbienti (l'Istituto autonomo case popolari). Ancora, queste organizzazioni hanno ruoli ben definiti e complementari tra loro e, secondo le varie norme regolatrici, debbono agire in modo congruo rispetto agli scopi assegnati e, soprattutto, hanno bisogno di risorse economiche per poter funzionare.

Naturalmente stanno sullo sfondo, come ha ricordato il relatore, senatore Pagliari, altri provvedimenti fondamentali per il cambiamento di paradigma della nostra pubblica amministrazione: ad esempio, l'azione amministrativa o il sistema dei controlli. o il sistema dei controlli. In particolare, nell'azione amministrativa abbiamo la necessità di superare una concezione profondamente stratificata nella nostra pubblica amministrazione: quella di privilegiare il formalismo degli atti come strumento per poter meglio rispondere all'esigenza di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione. In realtà, nel corso degli anni, tale approccio è degenerato, con varie inefficienze, prendendo il posto di quello che deve invece essere l'obiettivo dell'azione amministrativa, ossia il risultato al servizio dei cittadini e delle imprese. L'insieme delle organizzazioni che nel linguaggio quotidiano vengono individuate con l'espressione di amministrazioni pubbliche rappresenta, all'interno della Repubblica italiana, la parte numericamente preponderante sul resto e capillarmente e costantemente presente nella vita quotidiana dei cittadini. È ad essa che giorno per giorno si rivolgono il cittadino o l'impresa, per poter usufruire di quei servizi pubblici che rappresentano l'elemento fondante della nostra comunità. Il processo di riforma delle amministrazioni pubbliche ovvero di quell'insieme articolato di organizzazioni costantemente presenti nella nostra vita quotidiana, rappresenta quindi un passaggio fondamentale per la modernizzazione del nostro Paese o meglio, richiamando le parole del presidente della BCE Mario Draghi, una riforma di sistema con ampi potenziali di crescita per l'economia italiana, la cui attuazione può garantire una crescita del nostro prodotto interno lordo indispensabile per consentire all'Italia di rimanere ben agganciata Con la legge delega oggi in discussione si affronta il disegno organizzativo delle amministrazioni pubbliche, rendendolo predeterminato, stabile e certo. Conseguentemente, si agisce sull'entità dei mezzi patrimoniali e finanziari necessaria per poterlo far funzionare e sulle risorse umane, che con la loro opera al servizio degli apparati consentono al tutto di poter funzionare. Infine, si rinnovano gli strumenti giuridici ovvero sulle attività giuridicamente rilevanti, che consento alle amministrazioni pubbliche di raggiungere gli obiettivi propri attraverso schemi di comportamento legalmente precostituiti e coerenti con i tempi moderni. Ci sono molte norme che meritano di essere sottolineate, come ben ha fatto il senatore Pagliari nella sua relazione; mi limiterò a citarne alcune che mi sembrano molto importanti. Tra i tanti aspetti della riforma credo sia utile richiamare i punti salienti contenuti già nell'articolo 1, che introduce la cittadinanza digitale e che pone le premesse per un diverso rapporto tra cittadini e pubbliche amministrazioni, abbattendo le barriere fisiche dell'accesso alla pubblica amministrazione. Con i decreti delegati il Governo dovrà definire il livello minimo di qualità dei servizi *on line* assicurando a tutti i cittadini l'accesso Internet a tutti gli uffici pubblici, dalle scuole alle ASL; ridefinire il sistema pubblico di identità digitale volto a consentire l'accesso a qualunque servizio con un solo PIN, universalmente accettato in modo che il cittadino possa autenticarsi una sola volta presso uno dei gestori di identità digitale ed utilizzare tale autenticazione con qualunque erogatore di servizi *on line*, pubblico e privato, italiano e dell'Unione europea. Una vera rivoluzione. Si affronta in modo organico il problema della dirigenza pubblica con nuove regole per l'accesso e l'uscita. Si interviene sull'accesso alla dirigenza riconfermando il principio costituzionale dell'obbligo del concorso. I nuovi dirigenti delle amministrazioni pubbliche saranno i soli a dover rispondere della gestione e ci sarà un solo ruolo, niente più fasce; incarichi di massimo tre anni rinnovabili una sola volta. La contendibilità della dirigenza è indispensabile, come un ulteriore elemento che viene affrontato - cerco di concludere perché il tempo sta per scadere - con la legge delega è l'annoso problema delle società partecipate dello Stato, delle Regioni e degli enti territoriali che, come confermato anche dal rapporto Cottarelli, rappresenta uno degli aspetti più critici sul versante sia finanziario che organizzativo dell'intera amministrazione pubblica. Da questo punto un emendamento in questo senso - garantire al massimo la concorrenzialità e la contendibilità dei servizi pubblici locali, perché questo è un elemento che libera risorse, che dà opportunità di un migliore servizio a un minor costo per i cittadini. Si affronta inoltre con coraggio il tema del riordino, come dicevo, del sistema dei servizi pubblici locali, ed è da sottolineare la disciplina sulle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva, che fa chiarezza su tutte le attività che possono iniziare con una semplice comunicazione da parte dei privati e delle imprese, semplificando la vita ai cittadini, consentendo, quindi, di liberare quelle risorse e quelle energie di un nostro sistema di impresa che, nonostante l'arretratezza della pubblica amministrazione, è competitivo su tutti i mercati internazionali. Nell'ottica di questa riorganizzazione vi sono altre norme importanti di razionalizzazione e soppressione di uffici ministeriali, con funzioni che si sovrappongono a quelle delle *Authority* esistenti. Concludo con una citazione del professore Massimo Saverio Giannini, che già nel 1979 ammoniva il legislatore italiano ad intervenire ricordando che vi sono molte cause, talune anche assai lontane, che hanno concorso a produrre l'attuale situazione di grave disfunzionamento delle amministrazioni pubbliche, globalmente prese, e a suscitare per più parti di esse angoscianti preoccupazioni di ingovernabilità. Tuttavia, è opportuno in questo momento che di queste cause ci si occupi, onde non si ceda all'insidia di turbare il decidere disperdendosi per itinerari collaterali che potrebbero divenire recriminatori, ed oltre tutto quasi sempre sospetti di essere facili e gratuiti. Saggezza imporrebbe che si considerasse chiuso il passato e aperto il solo provvedere al futuro. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la possibilità di poter manifestare in quest'Aula il nostro forte disappunto per un provvedimento che porta con sé lo scioglimento di quel Corpo forestale dello Stato, così ha così ben illustrato nel suo intervento. Mi corre, però, anche l'obbligo di precisare meglio alcune valutazioni che in quest'Aula sono state fatte recentemente dal collega Giovanardi, quando, riferendosi all'antropizzazione delle nostre montagne in particolare, stabilisce che lì c'è un problema tra uomini e animali che va risolto a favore degli uomini e non a favore di un equilibrio e di una biodiversità che comprenda la convivenza più serena possibile tra uomini e animali.

di assicurare a quei piccoli Comuni, che sono le istituzioni organizzate sulle montagne, la capacità e la possibilità di garantire alcuni servizi. Nella politica dei tagli dei trasferimenti agli enti locali, infatti, sono proprio questi i Comuni che soffrono maggiormente, perché, nonostante il loro virtuosismo finanziario, non riescono più a garantire quel livello di servizi che negli anni passati ha reso più facile la vita nei loro territori. Vengo però subito al cuore della questione: nella nostra difesa del Corpo forestale dello Stato, c'è anche quella di un'idea di Paese e di territorio dove la convivenza tra uomini e animali è virtuosa e fruttuosa per tutti. Spesso dimentichiamo che, con il consumo di suolo del nostro Paese e con l'antropizzazione esasperata, abbiamo invaso il territorio che era degli animali, non viceversa. Da qui discendono spesso le tante polemiche, come quelle che abbiamo tristemente registrato nel caso

la cultura della convivenza tra uomo e animale in una coscienza unica della biodiversità che va garantita ai territori. In Europa ospitiamo il 30 per cento delle specie animali dell'intero continente ed il 50 per cento

intelligenti, che aiutino quelle comunità a mantenere il loro ruolo e la loro presenza su quei territori - il cui abbandono è senz'altro un grave rischio - ma secondo una coscienza moderna dell'equilibrio tra

L'indignazione che proviamo di fronte ad alcuni fenomeni che spesso salgono alla ribalta della cronaca, perché ci colpiscono con immagini cruente, la dice lunga: abbiamo una sensibilità ed un'attenzione a tutto questo,

quella struttura che le istituzioni hanno pensato tanti, tanti anni fa debba essere potenziata e rafforzata, non svilita ed assorbita in un ruolo magari solo amministrativo, che non ci aiuterebbe in quel percorso. Ascrivo al merito di Michela Vittoria Brambilla la capacità di portare all'interno della cultura del centrodestra il rispetto e l'amore per gli animali. Penso che ciò interpreti un sentimento diffuso, molto diffuso, tra milioni di cittadini e di elettori, che,

un provvedimento che delega il Governo ad affrontare questioni decisive, che andranno attenzionate dal Parlamento, valutando i tempi e i contenuti dei decreti delegati. altre norme di recente approvazione: penso in particolare a quella sui reati ambientali, che l'Assemblea ha approvato pochi giorni fa, introducendo quattro nuovi delitti colposi contro l'ambiente. Penso dunque che, sul testo in esame, in particolar modo con riferimento alla revisione e al possibile accorpamento del Corpo forestale dello Stato ad altri corpi di polizia, si debba fare molta attenzione, perché, nel momento in cui andiamo ad attuare un assetto normativo come quello modificato di recente, abbiamo la necessità che il nostro Paese si doti di un sistema di controlli efficace:

l'attività di prevenzione, oltre che quella di controllo e di repressione, non funzionerebbe. Occorre allora, sicuramente, una riorganizzazione delle funzioni in capo al Corpo forestale dello Stato, ma non un suo

al rapporto e agli accordi vigenti con il Ministero delle politiche agricole e con il Ministero

rispetto ai futuri decreti delegati. Abbiamo la necessità di costruire, nel nostro Paese, un sistema di polizia ambientale molto più efficace rispetto a quello che abbiamo oggi

al Corpo forestale dello Stato e le oltre 1.300 persone alle loro dipendenze, che svolgono un'attività importante, che è quasi autofinanziata, così come è quasi autofinanziato il funzionamento del Corpo forestale dello Stato, al netto ovviamente degli

che credo servirà a dare un indirizzo un po' più preciso, un po' più chiaro al Governo per la definizione delle funzioni, la sua riorganizzazione e soprattutto l'individuazione di un sistema nazionale di polizia ambientale che coinvolga, certo, le competenze di alta specializzazione che il Corpo è stato in grado di mettere a disposizione del nostro Paese, ma anche altri pezzi che svolgono funzioni analoghe: penso alle 2.800 unità di polizia provinciale che, ovviamente, possono integrarsi e intrecciare le loro attività e loro competenze; penso ai NOE dei Carabinieri e penso ad altri pezzi del nostro sistema che, in una diversa organizzazione, potrebbero anche costruire un argine molto più efficace contro i crimini La seconda considerazione che voglio fare, se mi rimane il tempo, riguarda gli articoli del provvedimento che vanno a sottolineare e a individuare la rotazione dei dirigenti e il rinnovamento del personale dirigenziale della pubblica amministrazione, mettendo a mettendo a disposizione dell'organo politico una maggiore responsabilità. Ecco: io credo che su questo occorra un'attenzione maggiore nell'applicazione della legge anticorruzione del 2011 che individuava nel segretario comunale un soggetto terzo in grado di di svolgere la funzione di verifica degli atti, ma anche di sovrintendere all'applicazione di questa norma. Credo che, da questo punto di vista, il provvedimento possa precisare meglio, con i decreti delegati, il ruolo di anticorruzione che anche la pubblica amministrazione deve svolgere all'interno dei singoli territori. Per questa ragione

Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, in queste ultime settimane l'ISIS ha moltiplicato ancora i suoi sforzi nella sua tanto vasta quanto folle politica del terrore, gli eventi al museo nazionale del Bardo a Tunisi, con le uccisioni di personale locale e di turisti, l'affiliazione di Boko Haram e Al Quaeda all'organizzazione del terrore e le brutalità perpetrate in Nord Africa. Alle barbarie nei confronti di bambini, donne e uomini si aggiunge la distruzione del patrimonio archeologico. Sono le molteplici e spaventose facce di una stessa medaglia. Circa un mese fa, dopo un intervento in Aula come quello odierno, incentrato sul patrimonio artistico e archeologico iracheno, ho redatto un'interrogazione cui molti dei miei colleghi hanno aderito e che dovrebbe ricevere risposta da parte del Ministro in Commissione esteri. Un breve aggiornamento, però, già si richiede, perché in queste poche settimane altri fatti incresciosi si sono verificati. Nonostante siano state smentite tramite analisi di immagini satellitari le apocalittiche distruzioni complete, tramite dinamite e *bulldozer*, dei siti di Nimrud, Khorsabad, Ninive e Hatra, tuttavia ingenti danni sono stati fatti e stanno per essere messi in atto in questi centri da parte del califfato. L'ultimo video in questa galleria dell'orrore

come per lo scempio compiuto al museo di Mosul, per distruggere mensole, cocci, maschere e statue che si erano conservate per più di 1.500 anni. Infine, le statue e le maschere di pietra poste troppo in alto sono state sfregiate da colpi di *kalashnikov* in modo che nulla che possa richiamare gli antichi idoli possa resistere nella memoria.

aveva importanza già allora, ma di settimana in settimana il suo valore, ahimè, sfortunatamente cresce e il pericolo è che aumenti ancora nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, a seguito degli interventi terroristici e di distruzione dell'ISIS. In conclusione, mi permetto di sollecitare la